Signor Presidente, chiedo scusa a lei, alle senatrici ed ai senatori, ma le Commissioni riunite 1a e 5a non hanno ancora terminato

approfondita, per quel che possiamo, tenuto conto che poi dobbiamo produrre un testo elaborato per l'Aula. Per questo motivo, signor Presidente, le chiediamo un rinvio dei

Presidente, io credo che ci siano dei momenti in cui va detta anche la verità, in quest'Aula. Prima il presidente Azzollini ci ha spiegato che sono stati presentati molti emendamenti.

male. Attenzione, perché state ripetendo le stesse cose che succedevano con il Governo Monti: rinvio della seduta, problemi di maggioranza, incapacità di trovare sintesi. Finisco chiedendovi: troverete questa soluzione? Non lo so. Ovviamente la soluzione vi serve per venire in Aula domani a dire che metterete la fiducia su un maxiemendamento

alla Presidenza da parte del prescritto numero di senatori la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, comma 1, sui disegni di legge nn. 356, 396, 406, 432,

in funzione di quello che purtroppo sta ancora succedendo nel mar Mediterraneo. Quotidianamente assistiamo ad una tragedia che si sta compiendo sotto i nostri occhi, ma ciò che ci sconcerta di più è che la tragedia si stia compiendo sotto gli occhi dell'Europa, mi sia concessa questa forzatura - ha le mani sporche di sangue. E non accettiamo i giudizi che sono

affinché questa tragedia, questa tratta di esseri umani, questa situazione scandalosa venga al più presto presa in considerazione dall'Europa intera. Il nostro Paese

assolutamente posizione su questa partita, mettendo a disposizione risorse economiche e, se necessario, anche risorse umane. Utilizziamo dunque

invaso, per così dire, le acque maltesi. Desidero segnalare questa modalità di operare molto incisiva, molto poco attenta e rispettosa, per quanto riferito, nei confronti di queste persone fatte immediatamente prigioniere:

e il nostro Paese, essendo assolutamente sproporzionato il raggio di mare di cui può fruire l'isola di Malta, che è certamente una piccolissima isola di fronte al nostro Paese. In secondo luogo, vorrei anche far notare che le associazioni dei pescatori siciliani da sempre si sono comportate in maniera seria, evitando il bracconaggio in mare e rispettando il mare, sia